**Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento,****su misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista e sistema nazionale di accoglienza dei migranti** è in corso la diretta televisiva della RAI. Passiamo alle interrogazioni sulle misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista.

la drammaticità della situazione e, parlando con la gente, tutti noi constatiamo quanto siano forti e pressanti la preoccupazione e la necessità di avere avere certezza della capacità delle Forze dell'ordine e del Governo di controllare il più possibile, nei limiti dell'umano, una situazione sicuramente di portata enormemente importante e forse, per certi versi, anche sovrastante le capacità complessive dell'uomo. In ogni caso, non bisogna mai arrendersi. Un tema forte viene fuori proprio dalle vicende francesi e,

prevenire il contrasto di natura religiosa e a garantire il massimo di tutela in una

sui giornali di oggi - e non è una novità - notizie di *leader* religiosi, di *imam* che vengono allontanati a seguito della scoperta del loro attivo impegno per fomentare la violenza, la guerra santa, atti di terrorismo.

e non risulta mai che vi siano state azioni di prevenzione. La domanda è dunque la seguente: c'è un'azione di prevenzione? In quei luoghi esistono controlli? Le Forze dell'ordine e le autorità fanno effettuare dei controlli perché ci possa essere davvero la prevenzione e si possano individuare i soggetti e le attività pericolose che da lì possono scaturire e spingere delle persone a compiere atti simili a quelli di cui abbiamo notizia in tutta Europa? Credo sia importante saperlo. Io sono dell'idea che i luoghi di culto debbano essere rispettati, ma certamente controllati,

Quali misure ha assunto per rafforzare la capacità operativa delle nostre Forze dell'ordine e, dunque, per prevenire e contrastare efficacemente il terrorismo di matrice fondamentalista? Al di là delle forze speciali, fondamentali ma non esaustive in questa lotta, ritiene che i nostri agenti siano preparati ad affrontare situazioni di emergenza terroristica? Il personale operativo è adeguatamente equipaggiato e in numero sufficiente a proteggere i tanti obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale? Ci risulta, dalla viva voce degli stessi agenti, dai segretari regionali del Sindacato autonomo di polizia (SAP), che, a dispetto di quanto lei racconta sui giornali, le nostre Forze dell'ordine versano in una condizione di "minorata difesa" rispetto non solo al rischio terroristico, ma anche ad altri eventi criminosi di minore pericolosità alcuni dati che lei certamente conosce: i nostri agenti si addestrano a sparare solo tre volte l'anno e spesso a loro spese; non vengono addestrati a sparare a obiettivi o sagome in movimento, né nelle ore notturne. E se un attentato avvenisse di notte? Le dotazioni sono obsolete,

In conclusione, signor Ministro, le chiediamo risposte certe. Non ci venga a parlare della percezione di sicurezza. Non vogliamo *slogan*. Vogliamo risposte certe e sicure.

che si sono caratterizzati per alcuni aspetti che vanno attentamente studiati. Essi hanno introdotto una nuova tipologia di reato di matrice terroristica, perché porta alla ribalta ed esalta la figura del cosiddetto attentatore solitario, e cioè colui che apparentemente non ha alcuna affiliazione diretta e quindi un collegamento preciso con una organizzazione terroristica, anche se poi dagli sviluppi delle indagini si rileva sempre una fonte di ispirazione o dei complici che aiutano il soggetto a compiere l'attentato. Si tratta di attentatori hanno, quasi tutti, disturbi mentali, in preda al delirio omicida in nome non si sa di quale dio, che purtroppo prendono di mira obiettivi cosiddetti civili e facili, quelli che in gergo vengono chiamati *soft target*, proprio perché aventi una scarsa capacità difensiva.

*(Misto-SI-SEL)*. Signor Ministro, gli atti terroristici collegati al fondamentalismo che stanno colpendo l'Europa, a partire dalla Francia, sono senza dubbio il risultato di molteplici cause. Certamente il ripetersi di questi episodi rappresenta anche il fallimento delle politiche di integrazione attuate da molti Paesi europei negli ultimi cinquant'anni. Coloro che compiono tali gesti sono, infatti, perlopiù immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in Europa e che evidentemente non si sono sentiti mai europei. Alla luce di ciò, chiediamo di sapere se questo Governo intenda lavorare seriamente a un programma di integrazione dei cittadini stranieri che riguardi gli elementi più importanti della vita sociale, a partire dal diritto di cittadinanza (il disegno di legge è fermo da troppo tempo in 1a Commissione al Senato), dalla formazione scolastica e dal diritto allo studio, dall'ingresso nel mondo del lavoro, dalla libertà di professare la propria religione in luoghi di culto adeguati e non in situazioni improvvisate. Non discriminare, e quindi garantire uguali diritti a tutti e tutte, è l'unico modo per non far crescere odio e radicalismo e garantire sicurezza. Il nostro Paese è meta relativamente recente del fenomeno dell'immigrazione, ma credo non debba fare l'errore di sottovalutare il tema dell'integrazione. Anzi, a nostro avviso, proprio la storia di oggi insegna che questo dovrebbe essere un elemento prioritario di intervento di un Governo che non guarda esclusivamente alle prossime elezioni, ma al futuro

a seguito degli eventi terroristici di matrice jihadista legati all'ISIS, è emersa nei consessi comunitari e internazionali, come quello della NATO, la necessità di incrementare l'alimentazione e l'uso delle banche dati europee e internazionali nei campi della sicurezza, degli spostamenti e della migrazione. L'*intelligence* basata su dati personali e biometrici diventa uno strumento fondamentale a perforare il muro di anonimato che ammanta il fenomeno del jihadismo e a corroborare il minuzioso lavoro di indagine necessario a smantellarne la struttura. Si rende, quindi, fondamentale una cornice intergovernativa integrata, capace di facilitare un approccio olistico all'acquisizione, raccolta e condivisione del materiale informativo da parte delle forze di polizia e militari. Le chiedo, signor Ministro, se non ritenga necessario svecchiare la normativa esistente e superare le compartimentazioni a tutt'oggi esistenti. Avendo dunque fisse le direttrici dettate dalla cornice internazionale di tutela dei diritti umani, la salvaguardia dell'interesse pubblico rilevante, la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica, lo svolgimento delle investigazioni difensive, le chiedo se non ritenga inoltre opportuno valutare l'ipotesi di una collaborazione tra i Ministeri dell'interno e della difesa, al fine di individuare una serie di casi in cui sia possibile rivedere le norme che regolano l'immissione di dati nel CED del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche con riferimento al trattamento di dati personali correlato alle operazioni militari svolte all'estero.

Ci sarebbe una lista di 14 nomi sospetti all'attenzione dell'antiterrorismo. Le chiedo di confermare se è vero che esiste un preoccupante filo jihadista che porta in Albania e che potrebbe comportare rischi anche per la nostra sicurezza interna. Il quesito principale che le pongo è, però, un altro. Il contrasto al califfato comporta una grande mobilitazione dell'*intelligence* - e i Servizi italiani stanno dimostrando di funzionare ma richiede anche e necessariamente la collaborazione dei musulmani che vivono in Italia, un milione e mezzo di fedeli ancora senza una legge che regolamenti le moschee. Esiste, e in che grado, questa collaborazione da parte soprattutto degli *imam* e da quanti di questi? Ancora, il Governo ha affermato il principio secondo cui si possono seguire nei confronti dei sospettati di terrorismo le stesse regole che si usano per i sospettati di mafia. Non ritiene opportuno prevedere per i *foreign fighter* che rientrano in Italia anche la fattispecie dei criminali di guerra per rafforzare questo tipo di prevenzione e repressione? Infine, lei ha invitato i poliziotti a portare con sé le armi di ordinanza anche fuori servizio. Il sindacato SAP ha replicato dicendo che le pistole sono troppo ingombranti per essere portate con gli abiti civili e chiedono, quindi, di potere comprare pistole più piccole con un porto d'arma diverso. Cosa risponde a questo tipo di problema?

evidenziati dalla stampa, ma anche dalle indagini di polizia - dei *killer* che hanno colpito a Nizza, che hanno colpito precedentemente a Parigi, o di quegli stessi di Bruxelles, attraverso il nostro Paese. Vede, Ministro, siamo sicuri che ci sia un'attività di *intelligence* importante, ma vogliamo avere la certezza che le nostre forze di polizia non siano mandate allo sbaraglio sulle strade dando ai cittadini una parvenza di sicurezza, sicurezza che, per le scarse strumentazioni a disposizione, non sono poi in grado di

in questo caso - gli idonei che non sono stati ancora assunti, poiché il concorso è stato bloccato. Lei sa benissimo che, se questo concorso non si sbloccherà, non si potrà procedere nemmeno al nuovo concorso previsto per il prossimo autunno. Ci chiediamo quali Forze dell'ordine abbiamo a disposizione sul campo,

a eccezione della parentesi di «Charlie Hebdo», dopo quel momento si è registrato negli ultimi mesi, e nelle ultime settimane in particolare così come rilevato prima dal senatore Mancuso - il fenomeno degli obiettivi più leggeri, i cosiddetti *soft target*, e della presenza di lupi solitari o emulatori, con devianze e problemi anche psichici. La prima domanda è proprio questa: come si intende procedere migliorando l'efficienza delle forze armate, delle forze di polizia e dei Servizi di *intelligence* rispetto a questo fenomeno, tenendo presente che i *soft target* - per esempio - nel periodo che stiamo vivendo, sono principalmente le località turistiche, i luoghi di grande affollamento - che non devono essere grandi come Nizza - ma anche tutte le località costiere che in questo momento sono interessate da flussi turistici?

Infine, per quanto riguarda le grandi organizzazioni terroristiche, vogliamo capire a livello normativo come il Governo vuole intervenire per

fare in quest'Assemblea è che il nostro momento storico ci consegna un contesto di sicurezza che esclude il rischio zero. Quindi, se l'obiettivo che ci si propone è azzerare il rischio, a mio avviso siamo fuori dal contesto di questo tempo. Noi Noi possiamo gioire ed essere orgogliosi dei risultati fin qui ottenuti, ma non possiamo negare che il rischio ci sia. Dunque, tutta la nostra attività è finalizzata a un solo obiettivo: comprimere il coefficiente di rischio. Noi lavoriamo per diminuire il rischio, nella consapevolezza che grandi democrazie occidentali, democrazie non occidentali e non democrazie, sono state colpite in ogni parte del mondo.

Se noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, dobbiamo dire la verità, e cioè che la prevenzione ha come obiettivo il non far verificare qualcosa: non realizzare un qualcosa, ma - lo ripeto - non far verificare qualcosa. Dunque, l'obiettivo che ci proponiamo ogni giorno è che non accada nulla.

perché non c'è alcun nesso matematico, scientifico, logico e causale che possa dimostrare che tutto quello che abbiamo fatto è la radice essenziale e il motivo unico per cui non si è verificato nulla.

Abbiamo arrestato 549 persone ed eseguito 2.859 perquisizioni su soggetti ritenuti contigui ad ambienti dell'estremismo religioso. Abbiamo indagato in stato di libertà 884 persone ed eseguito 102 espulsioni di soggetti evidenziatisi per il grado di radicalizzazione o per il sostegno ideologico alla jihad e 8 di questi provvedimenti hanno riguardato *imam*. Su questo argomento tornerò a breve, dopo aver detto - mi sono rifiutato di dirlo questa mattina in una conferenza stampa proprio per poterlo comunicare al Senato per riguardo a quest'Assemblea - che esattamente ieri è stato rimpatriato, essendo stato espulso per motivi di sicurezza nazionale, un marocchino di venticinque anni, Kachmat Najib, indagato per aver scaraventato per terra danneggiandolo, lo scorso 12 luglio, un crocifisso di legno all'interno della Chiesa di San Geremia,

anni, arrestato il 1° gennaio 2015 per il reato di danneggiamento aggravato per aver fatto irruzione nella chiesa di Cles, inveendo contro i fedeli e urlando espressioni di avversione alla religione cattolica. Il suo profilo di pericolosità è stato confermato da evidenze di *intelligence* che lo hanno indicato come inserito nella comunità islamica trentina e attestato su posizioni palesemente radicali. L'Arma dei carabinieri lo aveva già proposto per l'emissione del provvedimento di espulsione da parte del Ministro dell'interno per motivi di sicurezza dello Stato e, poi, è stato espulso per misure di sicurezza dall'autorità giudiziaria con un provvedimento dello scorso anno. A seguire, è stata eseguita

giusta e anche utile: ossia, separare sempre chi prega da chi spara. Un conto è la preghiera, un conto è l'assassinio in nome di un dio che non ha autorizzato quella preghiera. Il nostro lavoro sta nel rendere efficace questa separazione.

Altra cosa è il ragionamento sulle moschee. Noi stiamo avviando ancora un altro lavoro, che è la costituzione di un consiglio per le relazioni con l'Islam, dove siedono per la gran parte uomini di cultura e intellettuali italiani che hanno studiato il mondo arabo e l'Islam in Italia, e, contemporaneamente, abbiamo incontrato i vertici delle comunità musulmane in Italia. Dopo che questo consiglio per le relazioni con l'Islam ci ha fatto una proposta, li abbiamo fatti incontrare, sotto la mia presidenza, al Viminale. È venuta fuori l'ipotesi di realizzazione di un modello italiano di Islam che, ovviamente, non significa entrare nella dottrina di fede, ma significa dire basta agli *imam* fai di te; stop agli *imam* che arrivano in Italia avendo avuto una formazione radicale, e predicazione in italiano. E adesso stiamo lavorando per un qualcosa che sia condiviso dalle comunità musulmane,

che sono rigettati dalla comunità nazionale. Farli sentire fuori dalla comunità nazionale alimenta quel clima di odio che è poi l'*humus* per atti violenti.

delle norme. Prima di passare a questo argomento, però, io dico al senatore Malan che è vero che ci sono state segnalazioni dei fedeli. E noi plaudiamo

Se fossero più che sospettati, sarebbero o arrestati o espulsi per motivi di sicurezza nazionale. Mi sembra abbastanza evidente. Abbiamo svolto un lavoro assolutamente efficace anche da questo punto di vista.

il secondo attentato a Parigi del 2015: *soft target*, non un obiettivo sensibile, ma l'aggressione ai luoghi della nostra vita quotidiana. Cambia completamente il profilo.

numerose esercitazioni antiterrorismo. Lo abbiamo fatto in funzione del Giubileo, dell'Expo e degli altri eventi. Nell'essere assolutamente occupati

abbiamo ospitato un mese fa la finale di Champions e concluso l'anno scorso l'Expo. C'è stato un altro evento ai Fori l'altro ieri di grande importanza. Stiamo reggendo, quindi, anche alla pressione di eventi internazionali che abbiamo fin qui

polizia. Non tutti i presenti sono alla prima legislatura. Faccio appello a chi c'era nella precedente, ma anche questi tre anni non sono passati senza che la vostra memoria possa aver dimenticato quanto sto per dire.

Con quei soldi abbiamo fatto coriandoli? No: 300 milioni sono andati per gli 80 euro alle forze di polizia; 150 milioni - a breve il Consiglio dei ministri ne stabilirà la destinazione di merito

gli equipaggiamenti delle Forze dell'ordine. parlava della pista albanese. Noi ovviamente, per quanto riguarda la radicalizzazione, seguiamo tutte le piste. Non ci sfugge - è il motivo per cui abbiamo lavorato molto in quella zona - che quella è la vecchia rotta dei contrabbandieri e c'è il rischio che sia la rotta dei nuovi *foreign fighter*. La nostra attenzione è massima da questo punto di vista. Relativamente alle questioni che hanno riguardato le banche dati e quanto mi ero stato

le informazioni nell'ambito del sistema delle banche dati (in primo luogo europeo) e far sì che questo avvenga da parte di tutti i Paesi. Apparentemente ti spogli di un'informazione; nella sostanza, la versi in un contenitore dove troverai le informazioni degli altri e, quindi, saremo tutti più sicuri. Questa è una ragione per la quale, anche dal punto di vista della sicurezza,

continuare ad agire in tal senso, tenendo altissima l'attenzione e sapendo che in tutto questo c'è grande solidarietà, da parte di tutti gli italiani, verso coloro che hanno un compito così gravoso e importante. Signor Ministro, non siamo assolutamente soddisfatti, perché oggi non si parlava di un tema a piacere. Le ho posto delle domande specifiche, che sono agli atti, a cui la prego di rispondere, anche successivamente. Soltanto qualche piccolo chiarimento: le Forze dell'ordine sono in condizioni disastrose. Lei ha parlato di corpi speciali, ma si ricordi che a Nizza sono intervenuti i poliziotti e non le forze speciali. Ha parlato di finanziamenti: nella legge di stabilità erano stanziati 245 milioni di euro per la sicurezza interna. Ebbene, ben 112 milioni li avete spostati per per le missioni internazionali. Il Governo sta stanziando, proprio in questi giorni, ben 800 milioni di euro in armamenti. Quindi, i 150 milioni che lei dice di aver messo sulla *cyber security* sono ben poca roba. Questo atteggiamento non è assolutamente accettabile. Lei dimostra, ancora una volta, di non essere capace di svolgere il ruolo di Ministro dell'interno. Signor Ministro, siamo assolutamente soddisfatti delle sue risposte. Ci convincono le misure che il suo Ministero ha adottato e intende adottare per arginare i fenomeni in questione. Conveniamo sulla difficoltà di riuscire a contrastare attentati di questo tipo, spesso assolutamente imprevedibili, che confermano quanto lei ama giustamente ripetere e di cui ognuno di noi ha preso consapevolezza, e cioè che il rischio zero purtroppo non esiste. l'unico antidoto importante sia la prevenzione e mi pare di capire che su questo terreno, caro signor Ministro, l'Italia non sia seconda a nessuno. Ministro, noi non siamo assolutamente soddisfatti, perché non ha risposto alle nostre domande. Quindi, prendiamo atto del fatto che l'integrazione e la convivenza tra più culture non sono una priorità di questo Governo per prevenire il terrorismo. Sicuramente garantire il diritto alla libertà di professare la propria religione è importante,

da seguire per prevenire radicalismi e odio, e soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quella delle Forze dell'ordine.

a garantire la sicurezza di tutto il territorio nazionale, di tutti i siti e di tutte le stazioni: è pressoché impossibile. Proprio per questo è necessario impegnarsi

Lei ha detto giustamente che bisogna separare chi prega da chi spara. Bisogna però essere coscienti che esiste anche una zona grigia e ibrida, uscendo dall'equivoco dell'"islamicamente corretto" secondo cui i terroristi islamici sono nemici dell'Islam. Sono una costola impazzita dell'Islam, ma sono anche loro, purtroppo, Islam. E vedo nel mondo islamico ancora troppe contiguità, troppe ambiguità, troppe zone grigie sulle quali bisogna lavorare non solo dal punto di vista dell'*intelligence* e della prevenzione, ma anche dal punto di vista culturale. Se vinceremo questa sfida anche culturale, porremo le basi per vincere poi la battaglia contro l'ISIS. Ministro, l'enfasi con cui ha dato questa prima risposta non ci rassicura; anzi: troppo spesso, quando si mette grande enfasi nelle dichiarazioni, come lei ha fatto, si nasconde poi un vuoto operativo che ci preoccupa. La cosa che invece ci dà rassicurazione è la professionalità delle nostre Forze dell'ordine: ci sono uomini straordinari sulle strade, purtroppo spesso e volentieri

che i concorsi vengono fatti, che vengono assunti agenti delle Forze dell'ordine e soprattutto che c'è un lavoro di *intelligence* che impedisce l'ingresso nel Paese ai terroristi, perché questo è quanto è avvenuto con l'attentatore di Nizza e questo non deve accadere in un Paese che protegge i propri cittadini.

In questo senso inviterei, pur riconoscendo la grande professionalità delle forze di polizia, a innalzare ulteriormente il livello di attenzione sui luoghi della mobilità interna, perché uno degli aspetti che stanno emergendo in Italia

minori. Vorrei chiederle, signor Ministro, come si pone in questo contesto la previsione dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge enti locali che prevede, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, l'attivazione, affidata alla discrezionalità dei prefetti, di strutture ricettive temporanee con massimo 50 posti. vorrei sapere come si raccordano queste strutture con quelle di prima accoglienza già previste e cosa si pensa di fare per evitare rischi, in particolare che le nuove strutture di emergenza diventino permanenti, perché non è prevista una permanenza massima al loro interno. se non si procede, come immagino invece si stia facendo perché è previsto dal Piano per il 2016, ad adeguare tempestivamente e a potenziare il sistema ordinario di accoglienza, come si evita che questo diventi un binario parallelo di accoglienza e che si determini una concentrazione territoriale eccessiva di minori stranieri non accompagnati? In secondo luogo, secondo gli ultimi dati del Ministero del lavoro, a fronte di 12.241 minori stranieri non accompagnati presenti e censiti, ce ne sono 5.222 irreperibili.

oggetto di una serie di episodi, molti dei quali sono raccolti nel libro «Profugopoli» di Mario Giordano, dove si citano alcuni aspetti inquietanti. Non si tratta soltanto di casi di gravi inadempienze da parte di coloro che sono chiamati a

profughi. Si sa di moltissimi casi di persone stipate in ambienti dalle dimensioni non adatte, di persone che non vengono per nulla assistite quando invece le cooperative vengono pagate per assisterle,

esiste un'attenzione reale prima dell'assegnazione? Com'è possibile che si verifichino casi in cui avvengono nuove assegnazioni nei confronti di soggetti che sono già stati chiaramente segnalati e oggetto, anche in via definitiva, di provvedimenti? In questo ambito, voglio anch'io sollevare l'attenzione sui minori stranieri non accompagnati: purtroppo, in mancanza di una normativa specifica, sono affidati alle normative generali esistenti per questo settore, per i minori fuori fuori famiglia, normative assolutamente insufficienti e applicate in maniera preoccupante anche per i minori italiani. Il fatto che si siano perse le tracce di 5.000 minori stranieri è estremamente preoccupante e non paiono esserci misure

*(M5S)*. Signor Ministro, il Governo ha seriamente valutato i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale, al terrorismo interno e internazionale di natura fondamentalista, oltreché, soprattutto, la potenzialità destabilizzatrice del fenomeno migratorio che interessa il Paese tutto, soprattutto in relazione ai mezzi finanziari effettivamente stanziati? Sa, il Governo, sa lei, Ministro, che siamo in guerra, come ribadito dal Pontefice appena ieri? Sa che l'immigrazione può essere, quando non regolamentata, non governata, non trasformata da semplice accoglienza fisica in vera integrazione culturale e sociale, un'arma potenziale per le organizzazioni terroristiche? La Commissione europea, con specifico riferimento alla gestione italiana dei migranti, ha recentemente ribadito che «il numero di trasferimenti e di impegni rimane particolarmente basso se confrontato con il sempre maggior afflusso di migranti», rimarcando l'inadeguatezza degli organi preposti per la ricezione, l'identificazione e l'eventuale ricollocazione di immigrati in tempi certi e accettabili, così come descritto anche nell'ultima relazione della Commissione e che ci vede protagonisti di un rallentamento delle procedure che può essere disastroso in vista di un prevedibile incremento degli arrivi in Italia. Si chiede, dunque, cosa il Governo intenda fare al fine di: rendere rapido ed efficace il processo d'accettazione e di riconoscimento dei richiedenti asilo; coinvolgere gli altri Stati dell'Unione per una fattiva sinergia nel raggiungimento degli obiettivi posti dalla Commissione europea; di predisporre, con il supporto dell'Agenzia europea per la migrazione, le procedure di identificazione, gli eventuali ricollocamenti e rimpatri dei richiedenti asilo con tempistiche certe, oltre che rapide, e tabelle di marcia mensili e proporre la creazione di organismi specifici di controllo per l'impegno dei fondi stanziati a favore dei Paesi terzi, coniugandoli con piani di sviluppo locale, anche in relazione ai processi di democratizzazione dei Paesi di transito e di partenza, del rispetto dei diritti umani e del rispetto delle convenzioni internazionali; dotare le forze di pubblica sicurezza, cui si deve spesso riconoscere un impegno e una sensibilità sensibilità superiori a quanto stabilito dalla semplice osservanza del contratto di lavoro, delle necessarie risorse, d'organico e strumentali, per affrontare l'immane tragedia migratoria che investe il continente e, in particolar modo, il nostro Paese, magari dirottando mezzi finanziari che rappresentano attrattiva per operatori improvvisati cui sovente le prefetture concedono in affidamento diretto la gestione di Centri di accoglienza straordinaria (CAS) che successivamente risultano chiusi dalle prefetture stesse o, peggio, da procure della Repubblica.

Come sappiamo, oltre a un problema di assistenza molto sentito (almeno dalla nostra parte politica), c'è la necessità di una distribuzione di questi migranti anche in ossequio a un accordo europeo che prevede la presa incarico *pro quota* da parte di Stati membri. Al fine di raggiungere questo obiettivo è necessario che funzioni il primo anello di una catena, che è quello degli *hotspot* e, affinché il sistema che è stato progettato e ideato funzioni, non si può prescindere da un loro corretto funzionamento. Pertanto, organizzare al meglio il sistema degli *hotspot* è condizione essenziale per una rapida rapida identificazione con il sistema delle foto segnaletiche e delle impronte digitali e per il successivo smistamento verso i Paesi membri europei o per il rimpatrio, qualora ce ne siano le condizioni, che sappiamo essere regolate da

valide nell'impostazione delle procedure di intercettazione ed identificazione dei migranti, ma che stentano a funzionare nella maniera voluta e che potrebbero assolvere a una funzione diversa da quella desiderata e per cui sono stati concepiti. Signor Ministro, il sistema di accoglienza nel nostro Paese risulta essere particolarmente frammentato: un lato, abbiamo il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, gestito in collaborazione con i Comuni ed ANCI, che raccoglie circa 27.000 posti, dall'altro, il Centro di accoglienza straordinaria gestito dai prefetti, che riguarda circa 100.000 posti, ed infine i centri governativi, gli *hotspot*, in pratica gli ex centri di accoglienza per

che, perlopiù, riguardano l'accoglienza in grandi centri difficilmente integrabili nei tessuti sociali e territoriali, e che anzi rischiano di aumentare sentimenti di razzismo diffuso all'interno dei quali più facilmente si annidano fenomeni corruttivi nella gestione dei centri stessi. Alla luce di ciò, chiediamo al Ministro se e quando questo Governo abbia intenzione

del sistema SPRAR, a un percorso premiante di assegnazione di questi centri alla diretta gestione delle amministrazioni comunali. Infine, vorremmo conoscere quali sono le modalità di accertamento, da parte delle prefetture, di eventuali violazioni di diritti e di mala gestione dei centri governativi.

Il corto circuito che si verifica nell'accoglienza dei migranti è tutto europeo, nel senso che la *relocation* non sta funzionando, le cifre sono risibili (789 su 40.000, da quando fu emanata la direttiva europea), europea), con un numero crescente di richiedenti asilo che vorrebbero considerare l'Italia un Paese di transito e che poi sono costretti a rimanere qui, per cui abbiamo l'intasamento del sistema SPRAR

ma ci arrivano segnalazioni di identificazioni avvenute secondo l'approccio *hotspot* in altri luoghi: o direttamente sulle spiagge o nelle piazze di città. Le chiedo: in questi casi le procedure vengono seguite alla lettera o sono improvvisate? domanda è più importante: il Governo italiano si è battuto per superare la logica del primo approdo prevista dal Regolamento di Dublino III, che penalizza quasi esclusivamente l'Italia dopo l'accordo tra l'Unione europea e la Turchia, con la chiusura della rotta balcanica. Le chiedo: come giudica la proposta di riforma presentata il 4 maggio scorso dalla Commissione europea per rivedere il Regolamento di Dublino? È un passo avanti per l'Italia?

Ministro, nello scorso anno sono state valutate, da parte dei centri di identificazione e di espulsione,

è stato negato il diritto a restare, perché non ne ha: si tratta semplicemente di migranti economici. La questione è molto semplice, signor Ministro. Il suo Governo continua a mettere sulle spalle degli italiani i costi di mantenimento giornalieri, che in Italia ormai superano abbondantemente i 3 miliardi

quasi ci fosse un interesse sotto per mantenere il meccanismo di gestione dei clandestini sul nostro territorio. Concludo, Ministro, con un'ultima domanda: perché, a fronte delle espulsioni che poi non vengono effettuate, non istituite anche sezioni specializzate all'interno dei tribunali per dare velocemente la seconda valutazione e decidere, se il soggetto non ne ha dritto, di mandarlo al suo Paese?

fatto di chiaroscuri, in cui emerge abnegazione, come pure l'uso di numerosi mezzi e strutture pubbliche e private, come anche l'impiego di numerosi uomini e donne in divisa - cui va il nostro pensiero deferente nonché di migliaia di volontari dalla straordinaria sensibilità. Siamo in attesa di una modifica del Regolamento di Dublino, che forse non arriverà o comunque non accadrà nel breve termine; nel frattempo, l'apertura degli *hotspot*, così come così come il censimento attraverso le impronte digitali, che avrebbero dovuto snellire le procedure di accoglienza, procedono a rilento. In un mondo nel quale ha avuto un ruolo così importante Mafia Capitale, evidentemente se i centri di accoglienza non sono apparsi non sono apparsi trasparenti, o non sono stati mai controllati in questi anni oppure non c'è stato interesse a farli funzionare bene. Inoltre, tutto il sistema dell'identificazione e dell'espulsione dei migranti sta subendo l'impatto dell'accordo tra Turchia e Unione europea, che, con la chiusura della rotta dei Balcani occidentali, ha causato lo spostamento dei flussi verso l'Africa del Nord e quindi verso l'Italia. Come ritiene il Governo di iniziare a gestire, invece di subire, questi scenari inquietanti, in ossequio alla tutela dei diritti umani fondamentali, da intendersi non solo quelli

Augusta, ma anche sulle coste meridionali pugliesi, cittadini che soffrono le conseguenze della continua emergenza? Inoltre, poiché il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva il progetto della nuova guardia di frontiera e costiera europea, che riunisce l'agenzia comunitaria di frontiera Frontex e le autorità di gestione delle frontiere nazionali, la quale però non avrà effettivamente il potere di inviare forze in uno Stato membro senza un piano operativo, qual è la posizione del Governo a livello europeo su questa scelta, che comporta il rischio che il nuovo organismo sia privo del necessario potere per incidere in situazioni

Per rispondere a tutte le domande devo mettermi in modalità *tweet*. Ci provo, e spero di essere esaustivo. Poiché la senatrice Petraglia poco fa aveva ragione, nel senso che ho risposto solo parzialmente alla sua

in Italia ho voluto anche affermare esattamente la necessità di politiche che fossero di integrazione in quanto utili alla prevenzione della radicalizzazione. Quindi, l'integrazione serve anche sotto il profilo della sicurezza: più integrazione significa meno radicalizzazione e meno rischi di attentati.

i centri vengono ispezionati e monitorati dal punto di vista degli *standard* dell'accoglienza anche in partenariato con le organizzazioni internazionali, multilaterali e con quelle umanitarie, come l'Organizzazione internazionale dei migranti, l'Alto commissariato piena possibilità di accesso a tutte le strutture del nostro Paese. Voglio essere molto netto e chiaro. Noi abbiamo una linea, che è la linea italiana e la linea europea: tu scappi da una guerra o una persecuzione? Ti accogliamo. Tu non scappi da una guerra e sei migrante economico? Purtroppo non possiamo accoglierti e dobbiamo avviare le procedure di rimpatrio. Quando si parla di migranti economici, non si parla di terroristi.

Mazzoni. Abbiamo delle strutture dove prendiamo le impronte digitali e facciamo lo smistamento. Queste strutture si chiamano *hotspot*. Dall'*hotspot* il profugo esce identificato.

per proteggere le persone, sono stati circa il 40 per cento e quelli a cui le nostre Commissioni hanno dato il diniego sono circa il 60 per cento. I rapporti si sono invertiti, perché nel 2014 il rapporto era assolutamente capovolto. Cosa intendo dire? Che a livello europeo ci si dice

è difficile immaginare centri chiusi che, per anni e anni, debbano trattenere queste persone se non funziona il meccanismo dei rimpatri. Questo è il punto di collasso possibile della strategia europea. Noi ci stiamo battendo ma voglio essere molto chiaro: se voi chiedete al Governo di battersi in Europa per far pagare i costi della sorveglianza della frontiera, va bene; se chiedete a noi, come Governo, di batterci in Europa per sorvegliare quella frontiera con le navi europee, va bene; se chiedete di batterci per il ricollocamento dei profughi e perché questo funzioni, va Se però ci chiedete di far morire qualcuno in mare, questo non è il tipo di scelta che la democrazia italiana può sostenere. Noi salviamo tutti e, dopo, chiediamo con efficacia se sono profughi o migranti irregolari. Se sono migranti irregolari, li mettiamo mettiamo nel circuito del rimpatrio, se sono profughi no, in quanto li dobbiamo accogliere. Cosa voglio dire con questo meccanismo dell'accoglienza? Noi abbiamo un sistema che, evidentemente, spende delle risorse nell'accoglienza.

con la magistratura italiana e le prefetture fanno verifiche e controlli. Lavoriamo per evitare che ci siano ladrocini. Per quanto riguarda i punti deboli che sono diventati punti di forza,

non funzionava perché non c'era una struttura preorganizzata, in quanto il 2014 è arrivato due mesi e mezzo dopo la strage di Lampedusa, avvenuta ai primi di ottobre del 2013. Il secondo punto è che noi avevamo una ventina di commissioni per richiedere l'asilo.

da 20 a 50. E invece di fare come in un esame di maturità, con tutti i commissari che esaminano un solo migrante, abbiamo semplificato le procedure con esami *one-to-one*. Questo ha prodotto una straordinaria accelerazione del lavoro delle commissioni di asilo, che si è

L'altra questione, a proposito dell'Europa, è che noi eravamo l'emergenza europea. Se però dobbiamo essere onesti intellettualmente, come il dramma che stiamo affrontando ci chiede, non siamo più l'emergenza dell'Europa. Di fronte alla Germania, che l'anno scorso ha accolto

E non siamo né il primo, né il secondo, né il terzo Paese europeo, a maggior ragione visto in base alla popolazione. Dico poi al senatore Liuzzi che noi non abbiamo constatato l'enorme spostamento di flussi dalla rotta balcanica. E siamo contenti che ciò non sia avvenuto e che ci sia stato quell'accordo,

noi abbiamo i controlli delle prefetture, il controllo della magistratura e anche delle forme di partenariato per i controlli dell'Agenzia dell'anticorruzione. Se vi sono punti specifici e ulteriori oltre quelli citati nel libro, li segnali. È chiaro che le procedure di trasparenza sono degne delle nostre prefetture. Noi abbiamo un sistema di controllo efficiente. Poi, il ragionamento che ho fatto poco fa, del topo e del formaggio, appartiene a tutti gli investimenti che ci sono stati nel nostro Paese. Noi ancora paghiamo i conti di appalti che ci sono stati quindici anni fa, con processi di corruzione. Rispondo alla senatrice Guerra sul tema molto delicato dei minori non accompagnati. affaticano molto i nostri Comuni, soprattutto per quanto riguarda quelli siciliani. Il dramma, infatti, è nei Comuni siciliani, ed è inutile fare ragionamenti nazionali su questo argomento. La equa distribuzione ha funzionato, ma non vale

i minori stranieri non accompagnati sia cruciale, perché abbiamo tanti minori da sistemare quanti Comuni ci sono in Italia. Con uno a testa potremmo risolvere il problema. Mi sembra assolutamente corretta e importante la notazione che lei ha fatto, così come la sensibilità che ha mostrato rispetto al fatto che

conta episodi di siffatto genere. Basta citare il caso del Forteto, dove persone condannate per sevizie e violenze sessuali su minori si vedono affidare degli altri minori. Proprio per questo in tale settore occorrerebbe incidere molto profondamente.

Apprezzo tantissimo quanto ha detto in merito al fatto che una democrazia come quella italiana non possa accettare di far morire in mare in mare i richiedenti asilo per motivi economici. Ma voglio anche ricordare che, se avessimo speso la metà della metà di quanto è stato speso a livello europeo per salvare banche in cooperazione internazionale e misure di prevenzione, forse avremmo una situazione ben diversa. Non voglio citare il Forteto, ma non c'è solo la Sicilia per quanto riguarda i minori non accompagnati, ma c'è anche la Calabria. Voglio ricordare che tanti hanno scritto anche di traffico di organi... dal senatore Mancuso che avrebbero soltanto il compito di identificare e smistare i migranti. Purtroppo per debolezze del sistema che non dipendono solo da noi, ma anche da altri Stati, ci sono delle difficoltà a far funzionare al meglio Nonostante ciò, apprezzo lo sforzo che sta facendo il Governo soprattutto nelle città meridionali con il coinvolgimento dell'ANCI. E ritengo che tutto quello che si sta realizzando vada verso un miglioramento del sistema dell'accoglienza. Come italiani

che per noi è una vera e propria legge razziale in chiave moderna. Se non si cambia quella, il nostro sistema di accoglienza rimarrà variegato tra tutta la varietà di cui abbiamo parlato, dai CIE, ai centri di accoglienza straordinaria, ai centri per i richiedenti asilo. L'unico sistema che ha finora funzionato - come lei ci ha detto - è lo SPRAR. Io che vengo dalla Toscana ho esperienza diretta di cosa ha voluto significare l'accoglienza diffusa in tutti i Comuni, nei piccoli territori, con piccoli numeri, coinvolgendo non soltanto

Signor Ministro, mi permetto di insistere sul regolamento di Dublino. Capisco che riguarda solo in parte il suo Ministero, ma la riforma proposta dalla Commissione mantiene sostanzialmente invariata la gerarchia dei criteri di Dublino, riproduce gli stessi elementi fallimentari sui temporanei meccanismi di ricollocazione già in vigore, senza una ripartizione più equa delle responsabilità tra gli Stati membri. Credo che, se l'Italia non vince la battaglia fondamentale per una ripartizione più equa dei profughi,

La non risposta alle mie domande, signor Ministro, la dice lunga sulla volontà del Governo di affrontare seriamente la questione. Le ho chiesto perché non vengono aumentate le commissioni che devono valutare se i richiedenti asilo abbiamo o meno diritto, non mi ha risposto. Le ho chiesto perché non vengono istituite, all'interno dei tribunali, delle sezioni specializzate nel definire i ricorsi, affinché sia definito subito se uno ha diritto o meno e, nel secondo caso, sia rispedito a casa propria. C'è solo una soluzione: non vengano sul territorio nazionale, perché, nel momento in cui arrivano sul territorio nazionale, diventano oggetto di *business* e di E su questo il suo Governo ha una grande responsabilità, perché voi state scaricando gli italiani, che non hanno più assistenza sociale, e invece state mantenendo in albergo gente che è qui semplicemente senza averne diritto (il 60 per cento, lo dicono le statistiche).

senatore Liuzzi

Riconosco che, dal punto di vista dei controlli (a proposito dell'accenno al formaggio e ai topi), è importante che il Ministero abbia

condizioni di essere monitorati e controllati. La invito ovviamente ad accentuare siffatto tipo di sistema, sia per una sicurezza, sia perché su questo si gioca la credibilità degli aiuti internazionali.